dovrebbe così recitare: «Le stesse ordinanze riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009».

in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento

Chiediamo, signor Presidente, che il relatore e il Governo cambino idea sull'emendamento 1.309 (testo 2 corretto) perché, come lei può ben vedere, esso riguarda soltanto

*(PD)*. Signor Presidente, faccio un intervento in dichiarazione di voto sul primo subemendamento che viene in votazione e in discussione, il 3.5000/300, perché intendo porre anche in Aula il problema che abbiamo inutilmente proposto all'attenzione del Governo e della maggioranza in sede di Commissione bilancio. Molto rapidamente cerco di riassumere i termini della questione. Il testo originario del decreto, all'articolo 3, disponeva interventi a favore delle famiglie e delle imprese (ma in particolare delle famiglie) che avessero subito, non solo il danneggiamento, ma lesioni tali alla loro abitazione principale da rendere necessaria un'operazione di

al fine di realizzare l'intervento previsto dall'articolo 3 (in particolare dalla lettera *a)* del comma 1), si agiva, al di là delle somme rivenienti da aumenti di entrate disposte da questo stesso provvedimento, a valere sulle risorse del fondo strategico costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri utilizzando le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. Su questo fondo oggi, il Governo dice che sono disponibili fino a 7,5 miliardi di euro. L'articolo

costituito presso la Presidenza del Consiglio, utilizzando le somme del FAS. L'intervento è studiato in maniera che, come è scritto nella relazione tecnica,

dispone, in capo alle famiglie colpite dal terremoto, la costituzione del diritto soggettivo all'integrale ristoro delle somme spese

perché anche prima si disponeva in questo senso) è determinata «in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione,

Con mia somma sorpresa, e - credo - con l'umiliazione dell'intelligenza di tutti noi, il Governo pretende di sostenere che, pur disponendo diritti soggettivi che prima non c'erano e aumentando le provvidenze, la copertura può rimanere invariata.

lo stesso effetto dell'utilizzo dei fondi del FAS sul saldo netto da finanziare, sul fabbisogno, che è un dato di cassa, e sull'indebitamento. Ora, è del tutto evidente che ciò è tecnicamente impossibile, come del resto conferma lo stesso Governo presentando un emendamento che aumenta le risorse presenti in un fondo e che consente di rendere compatibili l'un saldo con l'altro. Per questa ragione, signor Presidente, in apertura della discussione su tutti i subemendamenti e sull'emendamento 3.5000/300, facciamo presente che, così stanti le cose, vi è una violazione evidente della norma di contabilità, un'arroganza del Governo, che pretende di non cambiare

Possiamo correre un rischio di tale portata su una calamità naturale che ha devastato un'intera Regione, mettendo a rischio la qualità e la quantità degli interventi a favore di quelle popolazioni? Credo che si stia commettendo un errore grave, intervengo per insistere affinché il Governo rinsavisca e non voglia umiliare la nostra intelligenza oltre che arrecare un danno all'intervento complessivo che si sta realizzando. Signor Presidente, la questione posta dal senatore Morando è di particolare interesse e rilievo e merita un commento, sia pure molto breve.

seppur dovendolo motivare meglio, ben avrebbe potuto quantificare il testo iniziale di gran lunga al di sotto di 4 miliardi, presumendo quindi che le modifiche rientrino comunque nei 4 miliardi complessivi. Ribadisco però che tutto ciò avrebbe potuto avere una motivazione migliore. Trattandosi di uno *spread* molto grande (tra 2 e 4 miliardi), è evidente che la modifica migliorativa per l'Abruzzo, introdotta dal lavoro in questo ramo del Parlamento, può situarsi all'interno di questo grande *spread*. Ciò nonostante, va sottolineato che le questioni poste sono di un certo rilievo ed è utile che il Governo rifletta su tale questione anche nel corso

l'emendamento 3.5000/300 è essenziale per caratterizzare e qualificare l'intero impianto del decreto n. 39 del 2009. Ciò per una questione di principio e di sostanza.

del Governo - nelle Regioni Marche e Umbria, con decreto-legge n. 6 del 1998, tutte le unità immobiliari furono considerate allo stesso livello per quanto riguarda la copertura integrale Non c'è stata alcuna distinzione tra abitazione principale e altre unità abitative, tant'è vero che in quel decreto, in diversi articoli, fu ribadito che le unità abitative riguardavano anche quelle a favore degli affittuari, a condizione che il proprietario si impegnasse a rilocarle alle stesse condizioni e agli stessi patti, e requisiti, anche le unità immobiliari adibite ad uso produttivo. È evidente che c'era una ragione, un principio ispiratore. Vengo alla sostanza del problema: noi veramente immaginiamo di poter procedere a un processo di ricostruzione pesante dell'Aquila capoluogo di Regione di una città in cui, all'interno dell'ampio centro storico, vi sono unità abitative pubbliche e private, e tra quelle private quelle adibite ad abitazione principale o a seconde case e a unità commerciali o artigianali

alla luce anche del fatto che c'è stato un chiarimento da parte della Ragioneria generale dello Stato sulla disponibilità dei fondi FAS.

Presidente, sull'emendamento 3.5000, che è fondamentale e centrale, sono già stati spesi gli argomenti che necessitavano dal collega Morando. Però a futura memoria, signor Presidente, signori del Governo e signori colleghi,

Questo ci dice il Governo: non aumentiamo i soldi per soddisfare questo diritto. Inoltre, questa mattina in Commissione bilancio la Ragioneria ci ha fatto presente che se non bastano i soldi non si fanno le altre cose.

contributo a fondo perduto per il finanziamento. Ora si mantiene il finanziamento agevolato, ma - vi abbiamo chiesto in Commissione - quale cittadino abruzzese, se ha diritto al 100 per cento di contributo, chiederà il prestito agevolato? Solo se è matto chiederà il prestito agevolato. Se lo farà, è perché gli diamo un contributo in conto interessi pari al contributo a fondo perduto per avere un mutuo superiore,

le parole senza senso e guardiamo alla sostanza: non stiamo garantendo un bel niente ai cittadini abruzzesi, rendetevene conto!

a sostegno delle loro aziende, con un 30 per cento da mettere immediatamente a disposizione di queste imprese. Si tratta di far ripartire alcune attività senza compromettere il conto generale, anzi, nell'emendamento suggeriamo una serie di di voci dalle quali recuperare questo costo di anticipazione. Si tratta però di un qualcosa di indispensabile, perché l'economia abruzzese non soltanto ha subìto una botta gigantesca con il terremoto, ma si trova adesso a subirne a cascata

apre una nuova finestra"), *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti sospesi, nonché gli ulteriori emendamenti e subemendamenti presentati, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, sugli emendamenti 2.800 e 3.5000. Esprime, quindi, parere di nulla osta, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui seguenti emendamenti: 9.0.10, a condizione che al comma 4 le parole: "sulle risorse iscritte nello stato di previsione del medesimo Dicastero per l'esercizio finanziario 2009, capitolo 7510, PG01" siano sostituite dalle seguenti: "sul Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio e smaltimento di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 28 dicembre 2007, n. 244"; a condizione che al comma 7, le parole: "nell'ambito delle risorse umane disponibili" siano sostituite dalle seguenti: "nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie"; 10.900, a condizione dell'approvazione del subemendamento 10.900/1; - 13.23 a condizione che sia infine inserito il seguente periodo: "All'attuazione della presente disposizione si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato"; 11.0.300 a condizione che sia infine inserito il seguente periodo: "All'attuazione della presente disposizione si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato". Esprime poi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 12.150. Esprime, infine, parere di nulla osta, sui restanti emendamenti e su tutti gli ulteriori emendamenti del relatore e relativi subemendamenti».

Signor Presidente, tutti - ritengo - condividiamo l'idea che la ripresa regolare dell'attività scolastica costituisca un elemento reale e simbolico di ritorno alla normalità, alla vita, e di ripresa delle prospettive di un futuro. Pertanto, i provvedimenti riguardanti la scuola sono decisivi e prioritari. L'emendamento 4.718, di cui sono prima firmataria, contiene alcune norme del personale della scuola e sulle strutture edilizie volte a garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2009-2010.

indicato - mettere in ruolo, coprendo tutti i posti disponibili, il personale docente e, per coloro che rimangono precari, deve essere confermato l'incarico per il prossimo anno. Vi sono inoltre norme che sostengono gli investimenti per la messa in sicurezza, la ristrutturazione e la costruzione di nuovi edifici scolastici. Si tratta di strutture permanenti, ma anche temporanee, che devono essere collocate vicino ai nuclei residenziali, anche provvisori. I essere spostati da una parte all'altra del territorio. Per questo sono previsti 500 milioni di euro per ciascuno dei tre anni 2009-2010-2011, regolarmente coperti. Segnalo infine la particolare negatività delle scelte scelte contenute nel decreto-legge del Governo per la scuola. Non si interviene sul personale e sulla stabilizzazione del personale docente e non docente. Le risorse che vengono destinate sono riferite agli attuali capitoli a disposizione del Ministero dell'istruzione che, sappiamo tutti, sono già assolutamente insufficienti ed inadeguati a coprire l'ordinario funzionamento scolastico. Sicuramente non hanno i finanziamenti necessari per l'assoluta straordinarietà degli interventi da realizzare

avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche e tramite la provincia relativamente agli uffici scolastici di competenza di questa.»;

visto che il G8 avrà una degna sistemazione a Coppito, quella può essere una sistemazione già data anche per far funzionare l'università a partire dall'inizio del prossimo anno accademico.

che affrontano un problema specifico dell'economia di quelle montagne. I due emendamenti, infatti, riguardano la zona del Gran Sasso e quella dell'Altopiano delle Rocche, che vivono sostanzialmente di turismo e di un'economia legata alle seconde case e che sono caratterizzati dalla presenza di piccoli centri abitati nei quali le persone sono rimaste - appunto - legate all'economia di quel territorio. Visto che si è deciso di non intervenire in modo sostanziale sulle seconde case, che sono un po' l'anima di quelle zone, chiediamo di intervenire sulle strutture turistiche. Infatti, se è vero che abbiamo un'emergenza in atto,

Dunque, se non si interviene subito con una programmazione adeguata, contribuiremo con la nostra disattenzione a spopolare ulteriormente quelle zone.

l'emergenza, in quelle zone e in quei Comuni che sono spesso abitati da poche centinaia di persone, bisogna ricostruire la speranza e il futuro. Se il Parlamento non lo fa e se continua a mostrarsi sordo, è evidente che i proclami sulla rinascita dell'Abruzzo e di quelle zone resteranno soltanto *spot* televisivi. televisivi. Chiediamo con forza che si prendano in considerazione questo bisogno e l'economia di queste piccole comunità.

la sospensione dei termini per i procedimenti pendenti avanti la corte d'appello d'Abruzzo. Sulla base dell'attuale formulazione

contenuta nella legge di conversione e non nel decreto-legge originariamente emanato, e quindi entrerà in vigore a giugno,

non si riescono ad estrarre ancora i fascicoli; bisogna ripristinarli e ripararli. Nel decreto non si stanzia un euro. Uno dei direttori del Ministero della giustizia si è recato in Abruzzo ad un'assemblea di avvocati e magistrati e ha ammesso di non avere

tutti gli emendamenti per facilitare l'approvazione del provvedimento, perché era assurdo che il decreto sul terremoto venisse approvato con un voto di fiducia.

delle persone che hanno avuto la sospensione dei tributi. Vi si chiede di concedere sei mesi di tempo agli istituti per comunicare ai cittadini quale sia il loro debito. Credo sia una norma di buon senso

L'INPS nega che i provvedimenti approvati da questo Parlamento, signor Sottosegretario, riguardino tutti i cittadini residenti in quelle parti del territorio colpite dalle calamità naturali, perché lega il beneficio della sospensione al danno;

del Presidente della Commissione lavoro abbiamo incontrato il presidente dell'INPS, che si è mostrato ampiamente disponibile; è stata emanata una circolare che ribadisce le stesse volontà e gli stessi comportamenti da parte dell'INPS: vengono escluse alcune persone residenti che lavorano altrove e così via. Ora non mi dilungo, non si fa altro che dare un'interpretazione autentica, trasferendo l'ordine del giorno che abbiamo approvato insieme in una norma di legge. Ditemi voi se il cittadino può andare dietro a comportamenti schizofrenici

vorrei sottolineare che, se si vogliono effettivamente aiutare imprenditori e professionisti operanti nelle zone colpite dal sisma, si devono prevedere misure che favoriscano il ripristino, nel minor tempo possibile, delle condizioni minime di operatività. Questi imprenditori devono poter insediare quanto prima la propria attività in nuovi locali, in sostituzione di quelli distrutti o danneggiati (soprattutto - e anche - se erano detenuti a titolo di locazione). L'emendamento si riferisce a questa fattispecie. Nel caso in cui i locali siano detenuti a titolo di locazione è importante intervenire per agevolare l'acquisto o la locazione tramite il finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato o, comunque, con indennizzi dedicati al reperimento di nuovi locali. Il credito di imposta non basta in questi casi, perché non si tratta di aiutare imprese operanti in condizioni di normalità ma che, magari, subiscono gli effetti di un periodo di recessione economica. Si tratta di imprese distrutte, in tutto o in parte, che devono ricostruire tutto daccapo, che devono trovare le risorse per riprendere la loro attività e quindi, prioritariamente, devono ripristinare i locali ove operano. Se, come fa questo decreto, si sospende o si differisce l'esecuzione di provvedimenti di rilascio per finita locazione, non possiamo non prendere in considerazione le condizioni di chi invece deteneva l'immobile in locazione per l'esercizio di un'impresa nel caso in cui questo immobile sia andato distrutto o, comunque, sia inagibile.

ma bisogna sapere che in quella Regione, colpita e distrutta dal sisma, molti paesi sono rinati grazie agli investimenti su quelle che vengono definite seconde case, ma che sono, in realtà, investimenti fatti da famiglie

alla desertificazione sociale di quelle zone: si può ricostruire il centro dell'Aquila, ma si rischia di far morire l'intera Regione. Questo è il senso importante e lo spirito dell'emendamento 6.705,

chiedono un differimento ed una ricontrattazione del piano di rientro del deficit sanitario. Signor Presidente, questo piano di rientro è stato sottoscritto dal Governo nazionale in un accordo del 2007, ed era riferito, nell'accordo a quel contesto economico, finanziario, demografico, socio economico, organizzativo e gestionale del sistema sanitario regionale. Credo che nessuno in quest'Aula abbia dubbi sul fatto che il contesto socio economico e sanitario della Regione Abruzzo sia mutato.

precari della pubblica amministrazione che operano nei servizi sociali, urbanistici e di assistenza, senza le quali si priverebbero le amministrazioni di personale importante in questa fase.

e, soprattutto, non si dà risposta a molti giovani.

servizio ai cittadini e alle imprese sul territorio. Per gli enti di secondo livello, e fra questi i consorzi di bonifica, è stata giustamente prevista la sospensione dei contributi da parte dei cittadini e delle imprese, salvo successiva restituzione. Questi enti, però, devono mantenere la propria attività e funzionalità

hanno ritenuto di chiedere al Parlamento e al Governo di modificare tale articolo. Il Governo, pur non volendo disattendere l'impegno assunto a finanziare le attività per la prevenzione del rischio sismico,

Questi volontari vivono solamente del 5 per mille: allora, poiché avevo presentato un emendamento e un ordine del giorno, chiedo al Governo un impegno.

della politica, ma dipendono dalla generosità e dalla volontà dei cittadini. Chiedo al rappresentante del Governo se può rispondermi.

indecente la scelta di cancellare dal decreto terremoto sostanzialmente l'articolo 11, che era quello sul programma di verifiche antisismiche, uno dei punti più positivi e innovativi dell'intero decreto. Le giustificazioni addotte dal senatore D'Alì sono - credo - in larga parte infondate. Se c'era un problema di coordinamento con le competenze delle Regioni, si poteva affrontare riformulando la norma. Ma perdere l'occasione del decreto terremoto per avviare un programma nazionale di interesse squisitamente nazionale che verifichi la sicurezza antisismica di quella gran parte di patrimonio immobiliare che si trova in aree ad alto rischio di terremoto credo sia un voltafaccia vergognoso, che contraddice peraltro

delle proposte di emendamento presentate dalla maggioranza e dal Governo più irricevibili tra tutte quelle oggi depositate.

un minuto del tempo dell'Aula, visto che stiamo votando e che il Parlamento è assolutamente impegnato nel lavoro, come ciascuno di noi può constatare, per leggere pochissime righe di agenzia di pochi minuti fa. Si tratta di una dichiarazione del presidente Berlusconi.

ma per snellire il Parlamento e arrivare a questo, ci sarà bisogno di un disegno di legge d'iniziativa popolare, perché non si può chiedere ai capponi» - quindi io e lei, senatore Cursi - «e ai tacchini» - analogamente - «di anticipare il Natale». L'ha detto all'Assemblea

C'era un'intesa con l'opposizione per concludere i lavori nella seduta antimeridiana, anche sforando l'orario delle ore 13. Abbiamo meno di 50 votazioni

subemendamenti sull'argomento. Ritengo che il subemendamento suddetto completi ed integri l'emendamento 10.900, che la Commissione ha approvato su istanza di tutti i Gruppi parlamentari, per l'istituzione di una zona franca urbana

della parte dell'impegno di bilancio relativo a un programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio, con l'emendamento proposto, per consentire alle imprese agricole abruzzesi di completare la realizzazione degli interventi previsti nel piano di sviluppo rurale, chiediamo al Governo che si faccia parte attiva perché venga prorogato di ulteriori 12 mesi il periodo di disimpegno automatico delle risorse impegnate in bilancio, sempre nell'ambito della programmazione regionale di sviluppo rurale. rurale. Signor Presidente, riteniamo che le risorse di sviluppo rurale diventano estremamente preziose e decisive affinché l'imprenditoria agricola abruzzese possa trovare il sostegno per ricominciare. Il comparto agricolo abruzzese ha qualità e caratteristiche altissime; è un comparto decisivo per l'intero sviluppo della Regione.

si debba riconsiderare, in accordo con le Regioni e le autorità europee, tempi, scadenze e condizioni. Questo è il senso dell'emendamento 10.240 e di altri che avevamo presentato si chiedeva di riammettere le domande di preadesione dei giovani agricoltori. L'emendamento 10.240 pone una questione specifica, ma vuole rappresentare in realtà la tematica più generale della rivisitazione dell'adeguamento dei piani di sviluppo rurale all'eccezionalità che si è creata. Stiamo parlando di risorse concrete, mirate alla competitività del settore, che possono fare molto per la prospettiva del settore agroalimentare della Regione. Rivolgo, dunque, un appello all'Assemblea affinché sostenga l'emendamento

momento che in interlocuzioni precedenti con i due rappresentanti del Governo mi si diceva che c'era stata la volontà di evitare l'attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, laddove fa riferimento alla riorganizzazione delle ex direzioni provinciali del Tesoro,

relativo all'impegno nei seguenti termini: «impegna il Governo a valutare con attenzione qualunque ipotesi di revisione territoriale degli uffici periferici del Ministero dell'economia e delle finanze».

una serie di misure che richiamano la ristrutturazione e la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze che attiene ad altre procedure e ad altri terreni di definizione, coinvolgendo maggiormente - come auspichiamo - le Commissioni competenti. Colgo Colgo l'occasione di questa dichiarazione di voto anche per apprezzare alcune modifiche che sono state introdotte sempre all'articolo 12, con l'emendamento 12.900 che abbiamo votato prima,

venga a proporre in Parlamento sul tema dei giochi una visione organica di riorganizzazione di questo settore così decisivo e importante per i suoi volumi finanziari, per gli interessi che coinvolge e per le persone che interessa come utenti e partecipanti ai giochi,

sarebbe necessario anche tenere conto delle patologie da gioco e di azioni di prevenzione e dissuasione di comportamenti che possono essere davvero molto negativi per quelle persone che sono indotte al gioco non solo per piacere, ma anche per forme di coinvolgimento e di sudditanza che rischiano di generare anche problematiche sociali di particolare rilievo.

un appello al Governo, al relatore e a tutti i colleghi,

un tempo e soprattutto risorse certe affinché si possano dare risposte ai cittadini abruzzesi.

che esso venga spostato prima, per dare assistenza a pazienti soprattutto anziani. Credo che ognuno di noi, se avesse la madre o una vecchia zia ricoverata in quelle condizioni, farebbe di tutto per poterla accudire nel modo migliore possibile. Di fatto quell'ospedale verrà comunque spostato: chiedo soltanto che venga spostato in anticipo per assistere i nostri concittadini. *(Applausi dai Gruppi PD e

intervengo soltanto per ribadire quanto abbiamo già più volte detto: il Fondo strategico per il Paese, dal quale sono state attinte le risorse da 2 a 4 miliardi di euro, dispone, per espressa dichiarazione del Governo, di un importo non impegnato pari a 7,5 miliardi di euro, per superare tutti i problemi di cui abbiamo parlato (prima casa, piccoli interventi e tutti gli altri interventi che sono stati richiamati). Vi abbiamo chiesto e vi chiediamo di elevare quella quota fino a 5 miliardi. Facciamolo, fatelo! Questo emendamento risponde a tale inderogabile esigenza. Solo in questo modo almeno una parte delle promesse che avete fatto agli abruzzesi potrà essere mantenuta.

**Il Senato non approva.**

Piacenza. Gli enti locali non riescono da soli a far fronte ai danni di vario tipo che sono intervenuti e quindi si chiede che il Governo intervenga prontamente per aiutare tali amministrazioni.

in fondo, il senso di riconciliare il Presidente del Consiglio con il Parlamento. Quando il Governo decise, con molti Ministri recalcitranti, di trasferire il G8 dalla Maddalena all'Aquila, il Presidente del Consiglio dichiarò che

senza toglierli alla Regione Sardegna che, nel frattempo, continuerà a realizzare tutte le opere infrastrutturali previste e programmate per l'originaria organizzazione del G8.

Presidente, credo sia l'ultima volta che possiamo insistere su questo argomento vorrei che i colleghi della maggioranza aprissero un po' le loro menti nell'immaginare...

nella universale ragionevolezza di questo provvedimento.

il dramma che ha colpito l'Abruzzo nella notte tra il 5 e il 6 aprile scorso ha distrutto non solo le case e i beni immobili, ma anche tante vite umane, ha dilaniato famiglie, ha lacerato un'intera comunità privandola dei suoi beni più preziosi: la casa e gli affetti. Al cospetto del dramma vissuto e che tuttora sta vivendo l'Abruzzo, la politica è chiamata a dare un segno di grande responsabilità e di unità per affrontare ed alleviare gli attuali disagi e avviare, quanto prima, una rapida ed efficace ricostruzione. E questo atteggiamento di responsabilità noi lo abbiamo dimostrato nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione e in Aula e lo dimostreremo anche oggi con il nostro voto finale di astensione. Un voto doveroso di solidarietà nei confronti delle popolazioni abruzzesi, pur non condividendo integralmente l'impostazione del provvedimento, rispetto al quale sono ancora forti le nostre perplessità. Esso è, infatti, un provvedimento monco; con esso ci si preoccupa giustamente di affrontare l'emergenza e di concorrere, grazie anche alla nostra sollecitazione, per intero alle spese necessarie per la sistemazione, la ricostruzione e l'acquisto della prima casa; ma la ricostruzione sarà e dovrà essere ben più articolata ed ampia. Questo provvedimento, infatti, non dà risposte rispetto alla necessità di recuperare un patrimonio immobiliare che è fatto non solo di prime case, ma di sedi di attività produttive, di seconde abitazioni, di un ampio patrimonio architettonico, di interi centri storici che devono essere ripristinati nella veste originale, come e dove erano, in quanto parte della storia abruzzese e dell'Italia intera. Questo patrimonio architettonico insieme alle seconde case rappresenta attrattiva e strumento per l'economia turistica del territorio abruzzese. Esso insiste anche al di là del cosiddetto cratere, su cui pare ci si concentri in modo quasi esclusivo. Cari colleghi, laddove c'è un nesso di causalità di causalità tra evento sismico e danno reale, diretto o indiretto, riteniamo lo Stato debba comunque intervenire a garanzia dei cittadini. Questo provvedimento purtroppo non è nelle condizioni di dare risposte al mondo produttivo abruzzese oggi in ginocchio. Non le dà alle piccole e alle medie imprese, ai laboratori artigianali, agli esercizi commerciali, ai professionisti in genere, ovvero a quei soggetti che lavorano e producono reddito in Abruzzo. Noi abbiamo formulato diverse proposte che sono contenute negli emendamenti presentati e purtroppo non accolti. Alcune di queste avrebbero garantito anche un introito di risorse finanziarie cui poter attingere. Rispetto al tema della copertura finanziaria di questo provvedimento, avremmo per la verità apprezzato una maggiore franchezza nel riconoscere l'esigua disponibilità delle risorse da mettere in campo. La ricostruzione graverà infatti pesantemente su tutti gli italiani - com'è giusto in parte che sia - dal momento che si attingerà ai fondi FAS, si ricorrerà alla razionalizzazione della spesa farmaceutica e del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, si ridurrà la dotazione del fondo per l'erogazione del cosiddetto *bonus* straordinario per le famiglie, per i lavoratori pensionati e non autosufficienti, nonché del fondo per la salvaguardia del potere d'acquisto delle famiglie. È chiaro quindi che non si tratta di nuove e diverse risorse, ma di tagli a risorse stanziate da precedenti provvedimenti anticrisi del Governo. E, laddove non si chiederanno sacrifici agli italiani, si provvederà mediante risorse presunte, frutto di successivi provvedimenti, che dovranno scaturire dalla lotta all'evasione fiscale e dal ricorso ai giochi, come se il terremoto d'Abruzzo fosse una nuova lotteria. Da qui le nostre maggiori perplessità. Rispetto a questi problemi noi abbiamo formulato proposte concrete, alcune delle quali accolte, come quelle relative all'istituzione di zone franche urbane nella Provincia dell'Aquila, all'integrale finanziamento delle prime case e al necessario coinvolgimento degli enti locali nella ricostruzione. Siamo però convinti della necessità

come pure ci pare ragionevole un prioritario coinvolgimento delle qualificate professionalità e delle risorse umane e strumentali locali, per garantire la qualità e la tempestività della ricostruzione, nonché il corretto impiego delle pubbliche risorse. Signor Presidente, particolare attenzione noi riteniamo che debba essere dimostrata alle attività produttive, commerciali e professionali in genere per una ripresa dell'economia locale che sta alla base della ricostruzione morale e civile di quei territori, così pure agli enti locali impegnati nel processo di ricostruzione. Tuttavia, nonostante la nostra piena volontà di dialogo, ribadita in quest'Aula, con il ritiro di gran parte dei nostri emendamenti, dobbiamo manifestare forti perplessità nei confronti del provvedimento in esame per le ragioni che abbiamo spiegato in precedenza. Possiamo quindi esprimere un voto di astensione, perché consideriamo questo provvedimento alla stregua di un primo importante intervento, ma solo di un primo intervento, al quale devono necessariamente seguirne altri.*(Applausi

e lo abbiamo dimostrato anche ieri in Aula con il ritiro responsabile di molti emendamenti - noi dell'Italia dei Valori abbiamo voluto, con le nostre proposte, esprimere la volontà di contribuire positivamente alle soluzioni più rapide ed efficaci. È infatti interesse di tutti ed è anche interesse di sane istituzioni, chiarire, correggere, migliorare, certo con l'urgenza che la situazione richiede, ma sapendo anche che la tragedia che ha colpito le nostre popolazioni avrebbe dovuto costringerci a riflettere meglio su molte cose. Per questo, signor Presidente, non condividiamo la definizione che da parti della maggioranza - e lo ha ribadito lo stesso presidente D'Alia - è stata data del decreto n. «Una rigorosa cornice dentro la quale si muoveranno le ordinanze». Con il nostro voto di astensione noi esprimeremo le molte perplessità sull'aggettivo «rigoroso», perché al contrario individuiamo molte indeterminatezze, ambiguità e confusioni, ma soprattutto esprimeremo le nostre molte preoccupazioni sul sostantivo «cornice», perché l'Abruzzo e con esso le famiglie, gli studenti, i lavoratori colpiti dalla tragedia, hanno bisogno se non di certezze, almeno di parità di diritti, di credibilità di risorse e di sicurezza dei tempi. Un primo elemento di debolezza è la non condivisa, anzi, contestata delimitazione dell'ambito territoriale di applicazione dei provvedimenti previsti dal decreto. Nessuno di noi vuole assalti alla diligenza, assistenzialismo di Stato o, peggio, resuscitare una sorta di Cassa per il Mezzogiorno *pro* terremoto: chiediamo semplicemente il riconoscimento che territori e intere comunità colpite dal sisma devono essere trattate con un uguale strumento normativo, che può e deve essere per tutti, sin da questa fase, una legge dello Stato. Un altro elemento discriminante che abbiamo voluto più volte riaffermare con le nostre proposte in Commissione e in Aula, è che il diritto di cittadinanza in Abruzzo non può valere di meno che in Umbria, Marche o Friuli ed è questo semplice principio che mette in discussione l'impianto stesso del decreto. Non solo in termini di princìpi ma di sostanza, noi chiediamo una equità, un pari trattamento, in parole semplici, l'applicazione di pari condizioni rispetto ad analoghe drammatiche situazioni che hanno colpito i cittadini italiani in precedenti esperienze. In quelle occasioni, signor Presidente, con il decreto-legge n. 6 del gennaio 1998, veniva consentito un contributo pari al costo di tutte le strutture, comprensivo di ogni adeguamento necessario al miglioramento sismico, rivolto non solo alle abitazioni principali, bensì a interventi mirati alla ricostruzione e al recupero di tutti gli immobili privati distrutti o danneggiati, quindi prime e seconde case, quindi anche immobili utilizzati per le attività produttive, industriali, commerciali, artigianali e quant'altro. Un elemento discriminante importante, perché non è pensabile (e si tradurrebbe negli anni in una ennesima presa in giro) progettare una ricostruzione armonica di un antico capoluogo di Regione ricco di storia immaginando la sua rinascita a pezzetti o a spezzatino. Nel corso dell'audizione in Commissione, il sottosegretario Bertolaso ci ha ricordato uno *slogan:* «Meglio avere operai in tenda, ma in grado di lavorare in fabbrica, piuttosto che operai in casa, ma con la fabbrica chiusa». Ebbene, il giudizio che noi esprimiamo sul decreto, per quanto riguarda gli aiuti alle imprese, non può essere affatto positivo. Alcune generiche misure annunciate sono condivisibili, ma mancano gli elementi base delle modalità attuative, gli importi massimali per singola impresa, i livelli di aiuto, la platea effettiva, lasciando le imprese in una situazione di grande indeterminatezza. Altro che ipotesi di rientro nell'Obiettivo 1 o di fiscalità virtuale di vantaggio, che rinvia molto opportunamente alle decisioni future della Commissione europea! Noi abbiamo chiesto un risarcimento completo per la ricostruzione di tutti gli immobili produttivi, come è stato fatto con il decreto-legge n. 6 del 1998, o un potenziamento degli ammortizzatori sociali per quei lavoratori privati interessati dalla crisi sismica e non rientrati nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, per i quali è necessario prevedere un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dalle disposizioni adottate per le Regioni